Signor Presidente, onorevoli senatori, «Evidente in generale è l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona». Queste sono le parole del presidente Napolitano al convegno «Giustizia in nome della legge e del popolo sovrano». Inutile dire che la pena, nel binario delimitato dalla sua funzione e dalla restrizione della libertà personale, non consente cedimenti rispetto a quegli ulteriori diritti e e a quegli ulteriori principi che sono sanciti dalla nostra Costituzione, quale ad esempio il diritto alla salute previsto dall'articolo 32. Il presidente Napolitano ha affermato altresì che «la politica, quale si esprime nel confronto pubblico e nella vita istituzionale, appare irrimediabilmente divisa, incapace di produrre scelte coraggiose, coerenti e condivise». Non mi nascondo la diversità che caratterizza il centrodestra e il centrosinistra nella visione globale del fenomeno giustizia e di quello carcerario; ciò nonostante, in considerazione della difficoltà del momento e della gravità della situazione carceraria, intendo qui evitare ogni contrapposizione, ogni tentazione di analisi comparativa: in una, ogni polemica. Intendo rappresentare la situazione per come essa è, esporre valutazioni in ordine ai dati oggettivamente emersi. Trovare con voi la soluzione ad una emergenza e aprire un discorso franco e sereno sulla possibile costruzione di un sistema normativo che disegni, forse per la prima volta, in sintonia con la Costituzione, cosa deve essere il carcere e come il carcere debba inserirsi nel più vasto e articolato mondo della giustizia. E se non vi devono essere cedimenti rispetto ai valori costituzionali, è doveroso fin da subito affermare che nel carcere deve essere assicurato l'ordine, deve essere garantita la salute e deve essere imposto, anche sotto il profilo logistico, il sereno svolgimento dell'espiazione della pena e della custodia cautelare. L'ordine, presidio del rispetto delle regole e ostacolo al formarsi delle sacche di anarchica confusione da cui originano la illegalità, la prevaricazione, la sottomissione degli uni agli altri, deve essere garantito da tutti gli operatori carcerari, direttori di carceri, educatori, polizia penitenziaria, ai quali tutti, indistintamente, va il nostro ringraziamento per la professionalità, l'abnegazione e l'umanità con cui quotidianamente adempiono ai loro doveri. E, al riguardo, non può non rilevarsi come, nonostante la recente integrazione di 820 unità, la scopertura di organico ammonti a 5.877 unità e come tale scopertura generi preoccupazione anche nel caso in cui - come si auspica - dovesse andare in porto l'assunzione di altre 1.611 unità per il 2012. Non è un caso, quindi, che, anche in adesione a specifica richiesta di organizzazione sindacale, si proseguirà nella strada già intrapresa di ridurre al minimo i comandi e i distacchi del personale della Polizia penitenziaria presso altre amministrazioni così restituendolo ai servizi di istituto, nonché di ridurre l'impiego del personale di Polizia penitenziaria nei servizi di scorta, a ciò aggiungendosi che l'enorme numero di traduzioni (185.755 nel 2010 per quasi 300.000 detenuti con un impiego di 769.000 unità di personale) e dei piantonamenti in ospedale aggrava vieppiù la scopertura dell'organico. Certo, anche le traduzioni rientrano tra i compiti di istituto. Ma è certo anche che se si modificasse l'articolo 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sì da rendere cogente che l'udienza di convalida avvenga in carcere e non presso l'ufficio giudiziario, ovvero si prevedesse che in caso di rito direttissimo l'arrestato o il fermato non transiti per il carcere ma resti nelle camere di sicurezza, ovvero ancora se la stessa procedura (arresto, convalida, direttissimo) fosse realizzata in modo più similare a quanto avviene nei Paesi con rito accusatorio, le traduzioni diminuirebbero vertiginosamente, e maggiore sarebbe la possibilità di utilizzare il personale della Polizia penitenziaria nel mondo del carcere. A seguito della riforma della medicina penitenziaria e della legge finanziaria 2008, si è realizzato il trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale. I rapporti tra carcere e ASL sono disciplinati da una serie di atti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il bilancio della riforma varia molto, a seconda delle realtà territoriali, con maggiori difficoltà di garanzia dei precedenti livelli di efficacia e continuità assistenziale medico-infermieristica nelle Regioni interessate ai piani di rientro debitorio. *Incidenter tantum:* dalla riforma deriva l'aumento del numero dei piantonamenti e del numero delle traduzioni ogni qualvolta (invero spesso) le ASL decidono di esternalizzare determinati servizi specialistici. Né posso tacere che, tra le Regioni a statuto speciale, la Sicilia, diversamente dalle altre, non ha adottato alcun intervento normativo per regolamentare il trasferimento delle funzioni sanitarie, con conseguente ricaduta di impegno sull'amministrazione penitenziaria che, per il solo esercizio del 2011 ha dovuto stanziare 12.400.000 euro per far fronte a quelle esigenze sanitarie che non le competono. Un'emergenza nell'emergenza penitenziaria è costituita dagli ospedali psichiatrici giudiziari e chiama in causa altri soggetti istituzionali che dovrebbero a pieno titolo farsi carico di un sistema che oggi offende la civiltà del diritto. L'insanabile contraddizione di una misura che si regge sul binomio carcere-manicomio gestita in luoghi che producono sofferenza, degrado, violazione della dignità e dei diritti fondamentali delle persone non può più essere tollerata in un Paese civile. Ancora oggi assistiamo alla odiosa sopravvivenza di questi luoghi che non curano, ma si limitano a contenere persone di cui nessuno vuole farsi carico, neanche quando è accertato il venir meno della pericolosità sociale che ne ha determinato l'internamento. La responsabilità della soluzione dello specifico problema penitenziario deve essere necessariamente condivisa con altri soggetti istituzionali giungendo alla completa sanitarizzazione, sul modello di Castiglione delle Stiviere, superando la presenza della Polizia penitenziaria, impegnata spesso in compiti non propri, e affidandone la completa gestione al Servizio sanitario nazionale. Nei giorni scorsi ho visionato il filmato realizzato dopo le ispezioni effettuate nei sei ospedali psichiatrici giudiziari, e non posso che condividere quanto scritto dal Presidente della Repubblica il 21 gennaio 2011, e cioè: «Ho così potuto prendere conoscenza di contesti igienico-sanitari e di vicende umane che hanno creato in me grande preoccupazione e profondo turbamento. Confido che non mancherete di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni misura amministrativa, organizzativa e legislativa idonea a consentire il superamento di situazioni che, in pochi casi, mi sono apparse assolutamente incompatibili con il più elementare rispetto della dignità delle persone e tali da integrare gravi violazioni di principi fondamentali della Costituzione». Una prima, concreta risposta a questo autorevole appello dovrà riguardare l'incredibile situazione dei 215 soggetti internati che permangono negli ospedali psichiatrici giudiziari, nonostante sia stata clinicamente accertata l'assenza di pericolosità sociale: una valutazione clinica cui non è seguita una analoga valutazione giuridica da parte del magistrato di sorveglianza, il quale, al contrario, ha ritenuto la sussistenza della pericolosità. E mi auguro che ciò, contrariamente a quanto taluno ipotizza, non derivi dalla mancata disponibilità degli enti locali all'idoneo riposizionamento del non più pericoloso. Bisognerà, altresì, pensare ad interventi legislativi finalizzati alla modifica dell'attuale sistema che consente, di fatto, la possibilità di applicare la misura di sicurezza *sine die,* indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato commesso. L'individuazione di un piano di trattamento sanitario con periodica rivalutazione potrebbe, ad esempio, consentire al giudice l'adozione di una misura analoga a quella prevista dall'articolo 286 del codice di procedura penale coinvolgendo *in primis* i dipartimenti di salute mentale. Così come potrebbero essere approfondite le soluzioni adottate in alcuni ordinamenti stranieri, quale quello spagnolo, che prevede un parallelismo tra la durata delle pene e la durata delle misure di sicurezza. Appare, inoltre, necessaria la creazione di strutture pubbliche di ricovero intermedio che, favorendo un più stretto raccordo tra magistratura e servizi psichiatrici territoriali,

A tal fine, potrebbe essere presa in considerazione la creazione di strutture di piccole dimensioni, facilmente individuabili sul territorio tra i piccoli ospedali soppressi o da sopprimere, con vantaggio anche per la completa regionalizzazione degli internati. Esprimo poi il mio apprezzamento per il lavoro della Commissione d'inchiesta, le cui conclusioni appaiono condivisibili. Con la stessa franchezza, devo però rilevare che l'adozione dello strumento del sequestro preventivo utilizzato per le strutture di Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino desta in me perplessità giuridica, mitigata solo dalla piena comprensione delle finalità che l'hanno determinata. Comunque, dando seguito ai provvedimenti emessi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, con decreto dell'agosto 2011 è stata istituita presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli la "sezione detenuti minorati psichici", si è provveduto ad effettuare lo sgombero delle zone detentive degli ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino e di Barcellona Pozzo di Gotto, si è attivato il procedimento di adeguamento ai rilievi mossi. Sul piano logistico, rilevante è stato l'intervento del Ministero, che ha provveduto nel triennio alla costruzione di 440 nuovi alla previsione di costruzione di 3.410 nuovi posti entro il 2013, alla ristrutturazione di 1.138 posti ed alla previsione di ristrutturazione di altri 710 posti sempre entro il 2013. Sono state, infine, aperte le strutture carcerarie di Rieti, Trento e Favignana ed è di prossima apertura quella di Gela, essendosi risolto il problema della condotta d'acqua. Il commissario delegato, infine, è impegnato nella rapida realizzazione della obsoleta struttura di Arghillà, monumento all'inefficienza del passato. A ciò deve aggiungersi che, in attuazione del piano carceri, sono state avviate le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori di 20 padiglioni aggiuntivi, per un totale di 4000 posti, con un impegno di spesa per 239 milioni di euro, lavori che saranno ultimati nel dicembre 2012. Altresì, previa riunione dell'apposito comitato di sorveglianza, si provvederà a varare, senza alcun danno per la sicurezza dei cittadini, il progetto di costruzione di carceri a bassa sicurezza per circa 5000 posti, in sostituzione degli 11 istituti penitenziari classici originariamente ipotizzati. I lavori saranno ultimati entro dicembre 2013, con un impegno di spesa di 349 milioni di euro. I 206 istituti penitenziari consentono una presenza regolamentare di 45.732 detenuti ed una tollerabile di 69.194 detenuti. Allo stato sono presenti negli istituti penitenziari 67.377 detenuti, ossia circa 2.000 in meno della soglia finale di tollerabilità.

sul totale, e il totale complessivo dei detenuti stranieri è del 36,10 tetto a cui si giunge nello spazio di tre anni (quattro anni fa il tetto dei detenuti stranieri era del 32 Di questo 36,10 per cento, 12.035 sono in attesa di giudizio e 12.147 in espiazione di pena: una percentuale questa davvero molto lontana dalle analoghe percentuali che caratterizzano la detenzione italiana. La tipologia dei reati all'origine della detenzione registra il primato dei reati contro il patrimonio, dei reati in materia di stupefacenti e dei reati contro la persona. Seguono i reati previsti dalla legge sulle armi e i reati contro la pubblica amministrazione. L'analisi dei dati consente di affermare che il tasso di crescita della popolazione detenuta è calcolabile in varie migliaia all'anno. Più precisamente, l'aumento è stato di circa 5.000 unità nell'anno 2009-2010 e di circa 2.500 unità nell'anno 2010-settembre 2011. Ciò si afferma in quanto, ai soli fini della valutazione del tasso di crescita, non può non calcolarsi il numero dei detenuti, circa 3.000, che nell'anno in corso hanno beneficiato della legge sulla detenzione domiciliare nell'ultimo anno di pena. L'analisi dei dati consente altresì di affermare che ogni anno si registra il transito in carcere di circa 90.000 detenuti provenienti dalla libertà (arresti in flagranza, fermo, custodia cautelare) e che di questi - mi rendo conto di affrontare

1.915 fino a 7 giorni, 5.816 fino ad un mese, 5.009 fino a 3 mesi e 9.829 fino a 6 mesi, per un totale di oltre 40.000 persone. persone. Va sottolineato che di questa aliquota di detenuti - come ho detto - la percentuale degli stranieri è superiore a quella degli italiani. I detenuti in custodia cautelare fino ad un mese ammontano nell'anno a 28.824, il che con tutta l'approssimazione del caso - equivale a dire che tale categoria di detenuti incide per circa 2.333 posti sul dato della presenza carceraria annuale. Quanto alle cause del sovraffollamento, non vi è dubbio che esse siano molteplici, sia pure con diversa significatività. L'analisi dei dati però consente, sia pure con molta prudenza, di escludere una particolare rilevanza delle norme introdotte nell'ultimo decennio a tutela delle esigenze di sicurezza dei cittadini. Infatti, quanto alle misure alternative e non omettendo di dire che il regime disegnato dalla cosiddetta legge Cirielli è stato in parte attenuato dalla legge del 2010 sulla detenzione domiciliare, si registra un aumento continuo di provvedimenti positivi sulle citate misure: gli affidamenti in prova sono passati da 1.818 del 2006 a 9.778 dell'agosto 2011; le semilibertà sono passate da 649 del 2006 a 921 dell'agosto del 2011; le detenzioni domiciliari (di cui all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario) sono passate da 1.618 del 2006 a 8.283 dell'agosto 2011. Il che, evidentemente, consente - se si vuole - un ulteriore approfondimento di ragionamento che per le conseguenze della legge Cirielli tali misure di libertà vanno verso soggetti quasi sempre incensurati o colpiti solo da una recidiva semplice e che scontano pene superiori ai tre anni, perché se fossero inferiori vi sarebbe la sospensione della pena fino a due anni prevista dalla legge Smuraglia o l'affidamento in prova al servizio sociale Analogamente, quanto alle misure dei cosiddetti pacchetti sicurezza, così come nella sostanza modificati dalla giurisprudenza europea, le incidenze sulla presenza carceraria sono limitate, peraltro con termini di non particolare significatività, e correlate a fattispecie criminose quali il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, il furto con strappo e il furto in abitazione, cioè a delitti che devono essere seriamente repressi, in ossequio alle ragioni di sicurezza dei cittadini. Se ciò è vero, e a me pare evidentemente vero, la riflessione sull'aumento della popolazione carceraria non può che incentrarsi su due specifiche cause:

Quanto alla presenza di detenuti stranieri, il cui aumento è speculare a quanto avviene in Spagna, Francia e Germania, evidentemente conseguenza dei flussi immigratori clandestini, non v'è dubbio che essa incida sul costante aumento della popolazione carceraria. Detti detenuti, infatti, ristretti in carcere per reati contro il patrimonio o attinenti agli stupefacenti o altro non essendo regolarmente presenti in Italia, non beneficiano di norma degli arresti domiciliari (non avendo trovato seguito quella giurisprudenza che immaginava come domicilio anche una panchina), o della liberazione e, per l'effetto, i processi a loro carico seguono le corsie privilegiate dei processi con detenuti ed arrivano rapidamente alla sentenza definitiva (così trasformando i detenuti in attesa di giudizio in condannati all'espiazione della pena). Giova altresì precisare che nei loro confronti è scarsamente applicabile e scarsamente applicata la misura dell'espulsione in sostituzione della pena detentiva sino a due anni; in ragione delle oggettive difficoltà dell'individuazione della loro provenienza geografica e della difficoltà di rendere operativi i patti di riammissione ove esistenti. Quanto alla custodia cautelare, i dati precedentemente forniti sui detenuti ristretti in carcere per brevi periodi (fino a un mese o tre mesi) denunciano inequivocabilmente come non sia puntualmente rispettato il criterio ordinamentale in base al quale la reclusione in carcere è una *extrema ratio*. Dubito che ciascuno di noi possa trovare un senso nella restrizione in carcere per tre giorni, per sette giorni, per dieci giorni, per quindici giorni o anche per 30 giorni. E, sia chiaro, anche per evitare inutili polemiche, quanto testé da me detto è ampiamente condiviso dal primo Presidente della Corte di cassazione, il quale ha invitato i magistrati «ad un uso sempre più prudente e misurato della misura cautelare restrittiva». A tacere di quanto affermato dal Presidente della Repubblica nel citato convegno, e cioè che si assiste a «un crescente ricorso alla custodia cautelare, abnorme estensione in concreto della carcerazione preventiva». Che fare quindi? Taluno, sulla cui buona fede non è lecito dubitare, immagina che la strada da percorrere sia quella, squisitamente parlamentare, dell'amnistia o dell'indulto.

che nel passato è sempre stata utilizzata come strumento emergenziale per risolvere un problema che non si voleva risolvere alla radice, sia per quanto concerne il mondo del carcere, sia per quanto riguarda il mondo della giustizia. Una strada che in passato ha sempre consentito al malato di respirare, ma che ha sempre rapidamente ricondotto il malato nel coma di partenza. Nel 2006, la presenza carceraria è scesa, in virtù dell'indulto, da 61.000 unità a 39.000 unità. Nulla è stato fatto per operare sul sistema, nulla è stato progettato negli specifici settori, e non è un caso che di lì a due anni la popolazione è andata a 55.000 presenze, per poi schizzare a 68.000 presenze nel 2010. Certo, siamo in presenza di un'emergenza e siamo costretti, quantomeno nell'immediatezza, a interventi tampone. La legge del 2010 sulla detenzione domiciliare nell'ultimo anno di pena, fortemente voluta dal ministro Alfano, ha avuto effetti positivi, consentendo l'uscita dal carcere a circa 3.000 persone, nessuna delle quali è poi evasa dalla propria abitazione. È una legge temporanea, la cui vita è limitata al dicembre 2013, data di ultimazione del piano carceri della positiva sperimentazione, potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento finalizzato alla sua eventuale estensione. Così come ulteriori approfondimenti meritano, con riguardo ai reati di minore gravità, l'attuale sistema della custodia cautelare e la stessa disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza: approfondimenti che tengano presente il concetto della restrizione in carcere come *extrema ratio*. Ma sono interventi tampone, non risolutivi o definitivi. Con ciò voglio dire che si deve aprire una stagione di sereno confronto tra le varie forze politiche, che abbia presente la necessità di definire un progetto globale di giustizia che porti la dovuta attenzione al sistema delle garanzie dei cittadini e che immagini il carcere come luogo di recupero, come luogo di cui interessarsi e non come luogo da esorcizzare, mettendo la testa sotto la sabbia come è d'uso per lo struzzo. In altri termini un progetto e un sistema che considerino l'edilizia carceraria solo come uno strumento logistico da modulare secondo l'obiettivo perseguito e non come la soluzione del problema, che abbiano ben chiari i valori della Costituzione e che abbiano la dovuta considerazione per i detenuti, non dimenticando mai che essi, indipendentemente dai loro misfatti, sono uomini e devono essere trattati come uomini. E come uomini possono essere assaliti dalla fragilità ed arrivare all'ultima scelta. Questo sarà il *vademecum,* nel settore, della mia azione di Ministro; sono certo che sarà anche il vostro. *(Applausi dai

di un malfunzionamento dell'impianto e dell'amministrazione della giustizia, su cui lei non si è voluto soffermare.

un epifenomeno macroscopico di un sistema della giustizia che non funziona. funziona. Salto il profilo dell'eccessiva durata dei procedimenti civili e penali, l'Italia ha riportato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 1.095 condanne,

in qualunque ordinamento democratico di ogni società. L'amministrazione della giustizia non è un settore come gli altri, ma è il pilastro su cui si fonda la credibilità istituzionale, lo Stato di diritto,

e per quanto riguarda omicidi, rapine, estorsioni e sequestri di persona la percentuale media degli autori che rimane impunita supera l'80 cento. Non c'è da stupirsi se poi un cittadino abbia, rispetto all'intero apparato della giustizia, una qualche resistenza, per non dire diffidenza. Né accenno qui al problema ancora più gigantesco dell'amministrazione della giustizia civile, sul quale spero si eserciteranno e approfondiranno altri colleghi. Il punto reale è che la giustizia civile sostanzialmente nel nostro Paese non esiste più: perché non ci si fa più ricorso, perché è troppo lunga, troppo lenta, troppo cara, troppo dispendiosa, e perché alla fine non si viene a capo di nulla. Tanto è vero

Onorevoli colleghi, 180.000 prescrizioni all'anno non rappresentano una vera e propria amnistia non regolamentata

cui stiamo assistendo drammaticamente nel nostro Paese? Questo mi porta ad affrontare subito il problema, non tanto dell'approfondimento che - mi auguro - verrà fatto da altri colleghi, ma

che coinvolge milioni di famiglie, la concessione di una vasta amnistia sia necessaria, urgente ed improcrastinabile. Di più: noi radicali riteniamo che l'amnistia sia l'unica soluzione possibile. Mi spiego: amnistia certo per i reati commessi da cittadini sottoposti a procedimenti penali, da detenuti in attesa di giudizio (lei ci ha ricordato da coloro che sono già sono stati condannati e hanno scontato una parte della pena. Ma onorevoli colleghi, signori del Governo, amnistia soprattutto per la Repubblica Repubblica - la repubblica del nostro Paese - costretta da anni a violare i principi fondamentali della nostra stessa legalità, le norme della nostra Costituzione, le nostre leggi, il rispetto dei diritti inviolabili della persona cui la vincolano i trattati internazionali, come dimostrano le sentenze. Insomma, noi viviamo in uno Stato fuorilegge, nel senso tecnico della parola; in uno Stato in flagranza di reato, ripeto, nel senso tecnico della parola.

perché come può assicurare in maniera credibile la sicurezza dei cittadini e perseguire con efficacia ogni forma di criminalità una Repubblica che, nell'esercitare questa funzione fondamentale, si pone essa stessa tecnicamente nella nella sistematica necessità di violare la legge? Lei, signor Ministro, ci ha detto - e molti ci dicono - che l'amnistia sarebbe solo una misura transitoria, destinata a svuotare le carceri per un breve periodo, e che è meglio la strada difficile, ma più efficace, delle depenalizzazioni di molti reati, la riforma delle norme sulla custodia cautelare. Io ribalto la discussione e le dico che l'amnistia è la precondizione, la premessa necessaria di qualsiasi riforma. voi oggi decidete di rinunciare all'amnistia, alla fine non avremo, come sempre, né l'amnistia né le riforme. C'è una tragica coazione a ripetere in questi argomenti e in queste convinzioni. Ricordo che, quando si discusse, nel 2006, in un dibattito che coinvolse il Parlamento, la proposta di amnistia e di indulto promossa dal ministro Mastella, per mancanza di coraggio alla fine si ebbe solo l'indulto, perché si disse che l'amnistia sarebbe arrivata dopo, al termine di un percorso riformatore che avrebbe avuto al centro l'emanazione del nuovo codice penale. Ricordo bene. E che ne è stato di quel codice penale, signori del Governo? Non lo trovate tra le riforme legislative della Repubblica. E per sapere quel che poteva essere e non è stato, bisogna andare in libreria e procurarsi il libro scritto a quattro mani da Nordio e da Pisapia, gli ultimi due presidenti nominati, uno dal Governo Berlusconi e l'altro dal Governo Prodi, della serie infinita di Commissioni incaricate di questa riforma, che non c'è, non è stata fatta e non è all'orizzonte. E intanto il tessuto del nostro diritto penale è stato lacerato da una serie infinita di interventi legislativi che non hanno più niente a che fare persino con quel codice, autoritario ma rigoroso, che pur ancora esiste. Insomma, una politica che si è rivelata inerte, incapace, che ricorre sempre a nuovi reati e nuove pene: ricorre al carcere come unica soluzione, senza nemmeno chiedersi se le strutture amministrative o penitenziarie siano in grado di assorbire i nuovi provvedimenti. Signor Ministro, onorevoli colleghi, la nostra richiesta, la nostra proposta di amnistia non nasce dal buonismo: nasce dall'intento di iniziare a governare un problema che scoppia e che è sotto agli occhi di tutti. Nasce dalla nostra concezione del diritto, che deve essere al contempo rigoroso e giusto; deve essere fondato su garanzie valide per tutti, e non sull'arbitrio o sul privilegio di casta o di classe. Amnistia, ne siamo convinti, come premessa delle riforme, perché se davvero riuscissimo per una volta a partire dall'amnistia, a concepire ed avviare una azione di governo per riorganizzare in maniera efficace e produttiva il lavoro giudiziario e la macchina della giustizia, allora sarebbe credibile, e possibile mobilitare il Parlamento e le Commissioni intorno ad un progetto di depenalizzazione, di decarcerizzazione, di limitazione della custodia cautelare, delle pene alternative al carcere. Signor Ministro, signori colleghi, a nostro avviso, non è possibile il contrario, e per due ragioni: in primo luogo, perché senza l'amnistia, senza una volontà politica determinata e un progetto politico di ampio respiro, ogni proposta le si sbriciolerebbe tra le mani, come accaduto al ministro Alfano (provi ad immaginare cosa accadrebbe all'interno della sua stessa maggioranza, se dovesse mettere mano alla Bossi-Fini o alla Fini-Giovanardi); luogo, perché, anche se per avventura lei riuscisse nel suo intento, gli effetti virtuosi e positivi dei suoi provvedimenti sarebbero fortemente limitati e, forse, in gran parte annullati dall'ingolfamento della macchina giudiziaria, dovuto all'impossibilità di smaltire milioni di processi pendenti. Quindi, il senso della nostra proposta - e spero sia chiaro - non è solamente il senso della amnistia come dato di attenzione ai diritti umani e civili dei carcerati. È anche e soprattutto una proposta di inizio di governo di un fenomeno. Infine, e per concludere, signor Presidente, spero che nella miseria della cronaca di questi giorni

e a renderci conto che, al di là dei miasmi insopportabili che escono un po' ovunque, da tutte le parti, esiste per noi parlamentari, finché saremo qui, la responsabilità parlamentare di contribuire alla soluzione e al governo dei problemi che il nostro Paese ha di fronte. È nostra responsabilità dare anche il segno e il simbolo di un'assunzione di responsabilità impopolare,

mi chiedo, penso, suggerisco e sono convinta che serva un tempo ulteriore di riflessione, e di dibattito aperto, fuori e dentro questo palazzo, un un dibattito che non si comprima affrettatamente oggi ma che lasci aperta la possibilità di qualche riflessione ulteriore. Presidente, che lei ha convocato una Conferenza dei Capigruppo per le ore 13 per l'organizzazione del dibattito. Ognuno si assume delle responsabilità. Mi permetto di avanzare la proposta a lei, signor Ministro, a voi, signori colleghi, che questo dibattito pure così importante, cui sono dedicate oggi due sedute, non si concluda stasera. Ci lasci il tempo della riflessione a tutti quanti quanti (è successo in altre occasioni molto meno importanti): si arrivi per lo meno alla settimana prossima, per riflettere meglio su cosa vogliamo, su cosa vogliamo, anche per gli agenti carcerari e per tutte le persone che intorno al carcere soffrono con i carcerati e vivono una vita quasi da carcerati. Mi permetto di chiedere a tutti, firmatari e non di questa convocazione, e a lei, signor Presidente, che si lasci a questo dibattito alto e nobile, rispetto a miserie che pure ci circondano e attanagliano, il tempo e lo spazio interiore

«La questione del sovraffollamento nelle carceri è un tema di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile». A sostenerlo è stato, con queste parole, il nostro presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo al recente convegno organizzato qui in Senato da Marco Pannella per indagare, esplorare e approfondire le problematiche inerenti il sistema penitenziario. In quell'occasione, il presidente Napolitano ha anche auspicato uno scatto dei politici per dare una risposta al dramma del sovraffollamento carcerario. Anche lei, signor presidente Schifani, si è espresso nello stesso senso, affermando, con la sua consueta chiarezza e determinazione, «Il sovraffollamento carcerario è un problema da affrontare con grande urgenza e nello spirito di coesione nazionale, che è indispensabile per ogni processo di riforma (...); anche per chi delinque valgono e vanno osservati sempre e e sopra ogni cosa i diritti fondamentali della nostra Costituzione». Infatti, non a caso l'Assemblea Costituente volle fissare in quel terzo comma dell'articolo 27 della Carta una concezione che che fosse in armonia con il principio della non afflittività della pena, ove recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Dal 2002 ad oggi - e soprattutto in questa legislatura, direi anche con risultati straordinari e inediti - con una serie di provvedimenti legislativi e di urgenza, il Parlamento e il Governo hanno inteso dare priorità al tema della sicurezza offrire ai cittadini segnali forti che fossero nella direzione di assicurare la certezza della pena; i risultati non sono mancati. Ammoderna un sistema di norme che non offra vie d'uscita in caso di recidiva e per i reati gravi, in particolare, dobbiamo convogliare ora, e bene, la nostra attenzione sullo stato i cui versano le nostre carceri. Sono ben consapevole dell'impegno profuso dal Governo nella delicata materia dell'emergenza carceraria e mi rendo conto che vanno individuati nuovi e più incisivi interventi che ne potenzino l'azione. Sono certo che una discussione matura, come è stato anche qui ricordato oggi, responsabile e libera da pregiudizi e da condizionamenti ideologici possa aiutarci a trovare quelle risposte a cui ci ha richiamato anche la Corte di giustizia europea, con una sentenza di qualche anno fa in favore di un detenuto che nel 2003 vi aveva fatto ricorso per le condizioni in cui era costretto a vivere la sua detenzione all'interno di una cella piccolissima, condivisa con troppe persone. Ancor prima, infatti, che un dovere della politica, ritengo che questa sia una vera e propria battaglia di civiltà che va combattuta fino in fondo per il bene collettivo. Un dovere di civiltà che, dopo la Corte di giustizia europea ci ricorda anche la recentissima sentenza del tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha riconosciuto il risarcimento pecuniario, pur modesto, ad un detenuto per danno esistenziale a seguito della permanenza in celle piccole, al limite della vivibilità, accogliendo le motivazioni dell'acuto e raffinato avvocato Alessandro Stomeo, propositore del ricorso; è un altro segnale che ci consegna la dottrina e che faremmo molto male a sottovalutare. Il tema della dignità della persona non è una prerogativa di questa o quella parte politica! Visito con regolarità gli istituti penitenziari e cerco di farmi un'idea costatando di persona le problematiche e le criticità: e sempre più mi convinco che in questo momento occorre davvero, senza speculazioni, senza partigianerie, senza prevaricazioni e senza strumentalizzazioni individuare percorsi condivisi e seri; piccoli passi in avanti ma che vadano nella direzione di dare un risposta concreta ai gravi e complessi problemi. Per tali ragioni ho accolto con grande convinzione l'invito della senatrice Bonino ad affrontare in maniera collaborativa la questione drammatica che ci vede qui oggi riuniti, e per la qual cosa desidero ringraziare anche il presidente Schifani. Il quadro emerso dalla visita alle strutture e dagli incontri con i detenuti e con gli agenti di polizia penitenziaria è tristemente desolante e suscita un senso di profonda indignazione, signora Presidente; un'indignazione che interroga la nostra coscienza di uomini ancor prima e ancor più che non la nostra responsabilità di parlamentari. Le condizioni di entrambe le carceri che ho visitato ad agosto scorso, quella di Bari e quella di Taranto, ad esempio, per il sovrafollamento esistente, per le gravi carenze strutturali per la inadeguatezza dell'organico sono incompatibili con il rispetto della dignità umana, con le finalità rieducative con la qualità del lavoro di quanti nei penitenziari, accanto ai detenuti, con grande spirito di servizio la propria opera e si impegnano lodevolmente ogni giorno, talvolta anche evitando il collasso del sistema. Questo è ciò che penso: chi vive la drammatica esperienza della detenzione e chi opera nei penitenziari merita attenzione; direi, merita un rispetto che sino ad oggi non è emerso in modo concreto ed efficace. Il grido di aiuto e di allarme non si leva solo dai detenuti ma anche dagli operatori del settore. Il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria rileva che le strutture detentive italiane si sono ridotte a meri depositi di vite umane: sono ben 11 le Regioni che hanno superato la capienza tollerabile; tra queste, la Puglia, perdurando una situazione di profonda difficoltà e di disagio vissuto sia dai detenuti sia dal personale penitenziario, anche quando questo è guidato da profili assolutamente autorevoli e dotato di grande competenza e professionalità, come accade nella mia Regione. I numeri, d'altronde, non possono indurre nessuno a girare la testa dall'altra parte, e fotografano una realtà drammatica che praticamente attraversa tutto lo Stivale. Come ha bene ricordato poc'anzi il ministro Palma, al 31 agosto, in Italia, a fronte di una capienza regolamentare di 45.647 posti, sono detenute 67.104 persone. I dati riferiti alla mia Regione, la Puglia, rendono ancora più evidente la situazione insostenibile: capienza regolamentare 2.458, detenuti presenti 4.490, praticamente il doppio. Va considerato poi che il personale di servizio, che deve fare i conti con turni di servizio, piantonamento, servizio di traduzione, riposi e assenze, è costituito sul territorio nazionale da poco più di 35.000 addetti: il rapporto non regge. In proposito, però, credo - lo dico con grande rispetto e prudenza - che dobbiamo forse disciplinare un po' meglio l'istituto del cosiddetto permesso sindacale, che deve lasciare categoricamente impregiudicato il diritto di rappresentanza, senza però che si lascino porte aperte a forme di abuso. Non credo che, in tempi soprattutto di rigore, non solo la sobrietà dei comportamenti, ma anche la corretta gestione delle sempre più inadeguate risorse economiche, possano consentire la presenza alle riunioni sindacali di ben tre persone per ogni sigla (in questo comparto ci sono oltre 10 sigle sindacali). Peraltro, vi è anche una disposizione, che riguarda l'accordo nazionale quadro del 2004 in materia di rappresentanza sindacale delle forze di polizia, che prevede il cosiddetto obbligo della consultazione

un po' di responsabilità da parte di tutti. La situazione è esplosiva anche sotto il profilo della sicurezza: come non ricordare anche oggi in questa sede che le reazioni di un essere umano costretto ad una situazione di degrado fisico e psicologico, al limite della esasperazione, possono degenerare nella violenza non solo verso gli altri, ma anche verso se stessi. Non può non colpire e lasciare indifferente il numero crescente di atti di autolesionismo e di suicidi: sono la spia di un disagio che va contro il tempo. Vanno dunque trovate strade nuove e risposte accettabili a problemi vecchi e ad emergenze nuove. Il Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931 non contemplava modalità di espiazione diverse dalla detenzione in carcere: la durata di pena era immodificabile, salvo la concessione della liberazione condizionale o della grazia, misure con il carattere di atto di clemenza, regolate dal codice penale. Con la Costituzione del 1948 venne introdotto il concetto di rieducazione; l'esecuzione della pena detentiva deve essere organizzata in modo tale da non rappresentare un'offesa per la dignità della persona e da consentire tutti quei trattamenti che appaiano più idonei al recupero sociale del detenuto. La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 va nella stessa direzione. Leggendo però il testo della raccomandazione e i principi elencati nella sua appendice si vede come le soluzione auspicate riguardano solo alcuni principi cardine cui si è ispirata l'attività di questo Governo e di questa maggioranza: il ricorso alla custodia cautelare, che tuttavia necessita di una riconsiderazione con possibili correzioni legislative ed anche una verifica delle procedure in sede applicativa (come peraltro ha autorevolmente ricordato di recente il primo presidente della Corte di cassazione); l'applicazione delle cosiddette misure alternative, la cui efficacia meriterebbe una maggiore attenzione da parte degli operatori; la finalità della pena detentiva; il rispetto della dignità delle persone. Il fenomeno non riguarda solo l'Italia. La crescita generalizzata della popolazione penitenziaria ha generato un grave sovraffollamento negli istituti penitenziari di tutta Europa. Il tasso di occupazione dello spazio carcerario

Nelle carceri dei Paesi dell'Unione si assiste ad una forte sovrarappresentazione dei migranti nella popolazione penitenziaria che in Italia supera il 35 I detenuti di nazionalità straniera sono particolarmente numerosi nei Paesi di recente immigrazione come l'Italia e la Grecia. Questo impone, quindi, anche un coordinamento che trovi un rilancio nelle attività diplomatiche, affinché le politiche migratorie siano coordinate con quelle penitenziarie, e una progressiva armonizzazione dei sistemi legislativi sovranazionali, con l'apertura di accordi bilaterali si ridisegni il sistema di funzionamento considerando la possibilità del rimpatrio per i cittadini stranieri per i quali è stata pronunciata una sentenza di condanna per reati commessi nel Paese ospitante. Non si tratta, infatti, soltanto di stanziare maggiori fondi, risorse economiche, soluzione peraltro in questo momento non particolarmente percorribile, ma anche di spingere l'acceleratore nel senso di una battaglia culturale e di civiltà che coinvolga tutti gli Stati membri e miri all'attuazione delle regole penitenziarie europee, sistema di principi lungimirante che prevede linee guida sia per la gestione dei detenuti che per la corretta gestione del personale delle carceri. Non occorre scomodare Voltaire,

e un nuovo modo di concepire la pena a cui si deve l'abolizione, nel mondo civile, della tortura e la riduzione del ricorso alla pena di morte. Oltre 250 anni fa, il marchese Beccaria evidenziava già come la pena non dovesse essere un sistema per «raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso», ma uno strumento per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro, ad opera dello stesso criminale o di qualcuno che dalla impunità di chi delinque potrebbe essere incoraggiato. La pena quindi, lungi dall'essere la rivisitazione di una forma tribale di vendetta, deve essere vissuta come un mezzo di difesa, un mezzo di prevenzione sociale. Siamo nel 2011 e percorsi di evoluzione nel senso di una civilizzazione della detenzione ne sono stati fatti in notevole quantità. Ora però bisogna compiere un ultimo reale e concreto sforzo in termini di qualità: l'ex ministro della giustizia Angelino Alfano prevede massicci interventi nella direzione dell'edilizia penitenziaria, senza trascurare il ricorso a misure deflattive e l'assunzione di nuovo personale. Tale piano prevede la realizzazione di padiglioni detentivi in ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi istituti penitenziari. È quanto mai opportuno accelerare in maniera prioritaria la procedura già avviata dal ministro Alfano di assunzione, nel complesso, di circa 2.000 nuovi agenti di Polizia penitenziaria, come peraltro previsto dalla recente legge 26 novembre 2010, n. 199. D'altra parte, anche la tenacia e la competenza del ministro Palma ci stanno già consegnando soluzioni percorribili e assolutamente condivisibili. Piano carceri, potenziamento degli organici polizia penitenziaria, depenalizzazione di alcuni reati e ricorso a misure alternative alla alla detenzione carceraria sono alcuni di essi: interventi indifferibili, tra l'altro auspicati e suggeriti anche dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, costituito in seno al Consiglio d'Europa. Dunque, l'impegno del Governo italiano c'è. Il mantenimento nella manovra finanziaria delle somme stanziate per l'edilizia carceraria ne è solo una testimonianza. E di questo va dato atto anche all'impegno del ministro Palma che ha sottratto con fondate motivazioni e con determinazione cospicue risorse all'incombente rischio di tagli. Ma anche le amministrazioni locali devono fare la propria parte. A Bari, ad esempio, c'è una perdurante, grave e inaccettabile situazione di stallo per quanto riguarda non solo il sistema carcerario, ma anche quello giudiziario nel suo complesso, costretto in uffici fatiscenti e, addirittura, inagibili da tempo, a causa

Sono frequenti i casi in cui, come accade in Puglia e a Bari, la burocrazia degli enti territoriali strozza le procedure amministrative sino a soffocarle nell'infausto destino del nulla e talvolta finanche dentro la opacità di un colpevole di un colpevole gioco di interessi, di potere e di personalismi su cui c'è ancora chi crede si possa costruire una carriera politica. La situazione a macchia di leopardo della gestione della medicina penitenziaria da parte delle ASL impone - come ha ricordato anche il ministro Palma oggi - una riflessione: occorre una maggiore volontà per superare l'attuale situazione di *impasse*, occorre concentrare l'attenzione sui tavoli regionali che coordinano l'attività delle varie Asl. La finanziaria per il 2008 ha stabilito il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, partendo dall'assunto che il servizio medico ed infermieristico di tanti operatori

nei penitenziari è di serie A? Vogliamo verificare quante risorse umane ed economiche (per non parlare dei rischi) si impegnano oggi per accompagnare i detenuti all'esterno dei penitenziari, negli ambulatori e negli ospedali pubblici, ogni volta che un servizio specialistico o un intervento ambulatoriale non può essere garantito all'interno dell'istituto penitenziario? Vogliamo accendere i riflettori su questo ed individuare delle soluzioni e delle ipotesi di miglioramento ad un problema che diventa dramma nella tragedia, dato che parliamo della salute di un soggetto detenuto? Lo scorso anno è stato compiuto un positivo passo in avanti per quanto riguarda l'applicazione dei protocolli sanitari. E' stato infatti avviato un progetto per la ridefinizione dei protocolli organizzativi relativi alla sanità carceraria:

alla società con meccanismi di inserimento agevolati; facendo in modo che le strutture penitenziarie divengano produttive di beni e servizi destinati all'interno e all'esterno, in modo da impegnare i detenuti ed avviarli ad attività la depenalizzazione di reati minori; riconsiderando le norme per la custodia cautelare a cui si ricorre talvolta in misura eccessiva, anche con riferimento a soggetti incensurati. riformare il codice di procedura penale, prevedendo che il giudice di merito decida per la condanna o l'assoluzione, demandando al giudice della esecuzione la quantificazione e l'identificazione della pena congrua, sulla scorta di una analisi

signor Ministro, onorevoli colleghi, la politica tutta deve sentire forte e pressante il dovere di dare una risposta rapida alle criticità di un settore che incrocia temi rilevanti di natura sociale, etica, economica e forse anche antropologica. Se accanto al tema dei costi della casta, ai cosiddetti privilegi, talvolta denunciati con enfasi e con una buona dose di demagogia, introducessimo nel dibattito che appassiona l'intero Paese, soprattutto in questi ultimi tempi, anche gli aspetti relativi alla credibilità, all'autorevolezza, alla responsabilità della classe politica e alla qualità del dibattito parlamentare e della produzione legislativa, forse accorceremmo la distanza siderale che separa

Signor Presidente del Senato, senatrici e senatori, signor Ministro della giustizia, membri del Governo, nel corso del suo intervento il Ministro ha voluto - e lo ringrazio per questo - dedicare una significativa riflessione alla situazione in cui versano gli ospedali psichiatrici giudiziari del nostro Paese, anche in relazione alle indagini svolte in materia dalla Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale. Avverto l'urgenza di spiegare il senso dell'articolata azione istituzionale, che è culminata nella unanime approvazione di una relazione scritta a questa Assemblea, nonché nell'adozione, anch'essa unanime, di provvedimenti coercitivi privi di precedenti nella storia repubblicana, provvedimenti coi quali, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, lo scorso 26 luglio è stato disposto, in relazione agli ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino e Barcellona Pozzo di Gotto, il sequestro, con ordine di sgombero immediato, delle stanze adibite alla pratiche di contenzione; il sequestro, con ordine di sgombero entro 30 giorni, delle celle caratterizzate da condizioni acute di criticità igienico-sanitaria e la conformazione integrale degli ospedali psichiatrici giudiziari - rispettivamente entro 15 e 180 giorni - alla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di incendio e dei requisiti minimi per le strutture psico-riabilitative. Naturalmente, la Commissione è consapevole di avere adottato dei provvedimenti eccezionali, esplorando l'articolo 82 della Costituzione fino ai suoi limiti estremi, ma si è assunta tale responsabilità a fronte di una situazione, accertata in sede di indagine, di vera e propria sospensione *de facto* della Costituzione repubblicana, una situazione che, come lei, signor Ministro, ha ricordato, ha turbato lo stesso Capo dello Stato, il quale, dopo avere preso visione del documentario realizzato attraverso sopralluoghi a sorpresa presso le strutture, ha parlato di "estremo orrore" e di situazione "incompatibile" con i principi della Costituzione repubblicana. Che cosa in concreto è emerso? La Commissione, nell'aprile del 2009, decise di avviare uno specifico filone d'inchiesta sulla salute mentale. Durante lo svolgimento di tale inchiesta, la Commissione ha ricevuto diverse segnalazioni in merito agli ospedali psichiatrici giudiziari e i relatori, senatori Saccomanno e Bosone, hanno suggerito lo svolgimento di ispezioni non annunciate presso tali strutture. Ciò che vedemmo - vi assicuro - destò in noi sconcerto, turbamento e profonda indignazione: celle luride, affollate al di là della soglia di umana tollerabilità; internati seminudi madidi di sudore a causa della temperatura torrida, per lo più sotto l'evidente effetto di forti dosi di psicofarmaci; servizi igienici in uno stato indescrivibile; penuria di agenti della polizia penitenziaria e pressoché totale assenza di medici psichiatri e psicologi; fatiscenza delle strutture, ai limiti - e talora oltre il limite - della agibilità; contenzioni in atto, adottate con metodiche inaccettabili e non refertate sugli appositi registri. Ai problemi cui ho fatto cenno deve aggiungersi, per Barcellona Pozzo di Gotto, la circostanza della mancata attuazione, nell'ambito della Regione Siciliana, della riforma della sanità penitenziaria, ciò che rende ancora più difficile - a detta degli stessi operatori - la situazione di quell'ospedale psichiatrico In sostanza, mentre per gli altri cinque ospedali psichiatrici giudiziari presenti nel nostro Paese vi è stata la devoluzione degli aspetti sanitari al Servizio sanitario nazionale, l'OPG siciliano dipende ancora *in toto* dal Ministero della giustizia, come il Ministro ha sottolineato questa mattina. dire che la Regione Siciliana non ha ancora recepito, a più di tre anni di distanza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2008. Riecheggiano ancora nella mia mente le parole con cui il relatore di maggioranza si rivolse alla Commissione, allorquando si trattò di riferire sugli esiti di quei primi sopralluoghi. Citando testualmente le sue parole dal resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 2010, «Durante il sopralluogo nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, la prima sede visitata, siamo accompagnati dalla vice direttrice. L'ospedale psichiatrico giudiziario è diviso in sei reparti. (...) Visitiamo per primo quello che è ritenuto il reparto più impegnativo in quanto dotato delle stanze predisposte per la coercizione. Al primo sguardo già appare grave il degrado igienico-sanitario. Chiarisco che questi termini non traducono il dramma delle condizioni in cui ci appaiono pareti, pavimenti, bagni, letti, effetti letterecci che vengono cambiati ogni 15 giorni (se è possibile) ed indumenti medesimi dei detenuti. Nelle due stanze predisposte alla contenzione c'è un paziente detenuto scarsamente sedato (perché in grado di rispondere), coperto da un lenzuolo ma completamente nudo, con polsi e caviglie strettamente legati agli assi metallici del letto; non può articolare nemmeno minimamente gli arti. Il letto, oltre che arrugginito, è predisposto con un foro centrale per feci ed urine a caduta libera in una pozzetta posta in corrispondenza sul pavimento. Quel foro centrale era arrugginito per il passaggio di feci ed urine di tanti pazienti che lo avevano preceduto negli anni. Non c'è alcuna idea di salute né tentativo di cura ma abbandono, deposito di umanità traviate senza prospettiva: un'incuria disumana. Questa è la mia sensazione». Ho voluto citare testualmente le parole del relatore di maggioranza, all'indomani dei primi sopralluoghi, non certo perché quelle del relatore di minoranza siano state meno pregevoli o incisive, ma per dimostrare l'*idem* sentire delle forze politiche di fronte alla situazione di incostituzionalità di fatto che abbiamo purtroppo accertato. Le risultanze delle articolate e prolungate attività d'indagine svolte sono ora, letteralmente, sotto gli occhi di tutti: il documentario, dopo essere stato parzialmente veicolato dalla trasmissione «Presa diretta» su RAI 3, è adesso integralmente visibile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica. Nel corso delle indagini abbiamo accertato che in molti casi, con una prassi che non saprei come definire se non *extra ordinem*, le misure di sicurezza di ricovero in OPG vengono prorogate anche a soggetti che hanno perduto, in tutto o in parte, la pericolosità sociale; ciò per la ragione che il magistrato, in assenza di un progetto terapeutico e di una presa in carico da parte del competente dipartimento di salute mentale (ossia le ASL), preferisce prorogare la misura. Sul punto trovo opportuno citare il brano di un'audizione in Commissione di inchiesta. A parlare è un magistrato di sorveglianza che afferma quanto segue: «È in questo che consistono le proroghe in deroga, anche dette ergastoli bianchi. Fino a quando qualcuno fuori non si assume la responsabilità di controllarli, diciamo che stanno meglio dentro che fuori. Questa è la situazione». La brutalità di tale ragionamento è evidente a tutti, ma vorrei che vi soffermaste a pensare che, quando si parla «proroghe in deroga», si nasconde, dietro a un tecnicismo giuridico, una prassi di sistematica lesione di disposizioni costituzionali, quali gli articoli 2, 13 e 25 che tutelano la libertà personale e l'articolo 32 che tutela la salute come fondamentale diritto della persona. A tale riguardo, quando in sede di audizione chiesi ad un altro autorevole magistrato, presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, di prendere posizione sulla conformità alla Costituzione di tali prassi, questi rispose testualmente: «Non possono trovare nessun fondamento nell'attuale ordinamento». Dovete infatti considerare che, con la proroga *extra ordinem*, una persona non più socialmente pericolosa viene a essere, nel contempo, privata della libertà personale e del diritto alle cure, senza un valido titolo giuridico. 1.500 internati, quasi 400 sarebbero dimissibili perché non più pericolosi socialmente. La Commissione non si è peraltro limitata a registrare le suddette criticità e a far emergere un'area di incostituzionalità di fatto: a fronte della descritta situazione, ha individuato una serie di possibili interventi correttivi, in parte realizzabili a legislazione invariata, in parte richiedenti una attività riformatrice. A legislazione invariata occorrono: interventi urgenti di revisione e adeguamento dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli arredi sanitari agli *standard* ospedalieri attualmente in vigore a livello nazionale e regionale; l'introduzione di una nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria, che sia conforme ai piani sanitari regionali della salute mentale delle Regioni sede di OPG; un più stretto raccordo tra magistratura e servizi psichiatrici territoriali, nonché l'elaborazione di linee guida funzionali ad agevolare un più frequente ed omogeneo ricorso alle misure alternative all'internamento; una rivalutazione sanitaria specialistica dei singoli casi, uno ad uno, finalizzata all'elaborazione di un progetto riabilitativo individuale di recupero psicosociale, dettagliato per tempi, luoghi, tipologie di intervento e obiettivi perseguibili e soggetto a verifiche periodiche di attuazione e avanzamento; recepimento urgente della riforma della sanità penitenziaria da parte della Regione Siciliana; creazione di strutture pubbliche di ricovero intermedio, che possano rappresentare una adeguata alternativa alla scelta tra internamento in OPG e ricorso a modalità di libertà vigilata non sufficientemente sicure. vanno segnalati due possibili livelli di intervento legislativo, enucleati in sede di relazione scritta a questa Assemblea: una riforma radicale e di sistema, che importi una abolizione dell'istituto della non imputabilità per vizio di mente; ovvero, interventi di modifica mirati, volti a eliminare chirurgicamente alcune delle criticità più manifeste della legislazione vigente (come l'abolizione delle misure di sicurezza provvisorie, l'introduzione della necessità di valutazione collegiale della infermità mentale e della pericolosità sociale e l'introduzione del principio di parallelismo fra durata della pena e durata della misura di sicurezza).

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, a febbraio 2010 approvammo in quest'Aula

questioni molto concrete, e chi ha visitato le carceri lo sa. Ci sono delle sezioni di alcune carceri storiche del nostro Paese nelle quali persone di minore pericolosità possono avere, da parte delle forze preposte,

La sanità penitenziaria è una delle riforme, secondo me una di quelle buone, che sono state fatte e dalle quali, come parlamentari ma anche come cittadini italiani, dovremmo cercare di imparare

va avanti sull'abnegazione del personale, dei volontari nonché della Polizia penitenziaria; l'assistenza ai singoli che hanno problemi, come l'HIV o altre situazioni invalidanti, spesso avviene grazie alla singola guardia di Polizia penitenziaria che si muove a compassione però, non è accettabile perché evidentemente procura problemi dal punto di vista organizzativo. È necessaria, poi, una maggiore programmazione da parte delle ASL: cosa ci vuole per sapere che alcuni medicinali non possono essere richiesti giorno per giorno da un'istituzione come il carcere, che è aperta 365 giorni

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io sono tra i firmatari della lettera con la richiesta di questa seduta straordinaria del Senato, perché sono convinta della necessità di di misure immediate e straordinarie per affrontare l'attuale emergenza carceraria del nostro Paese. Appartengo inoltre a quella ampia schiera di senatori che hanno presentato in questa legislatura numerose interrogazioni su tale argomento; in esse venivano stigmatizzati i dati di carattere generale, ma ognuno di noi ha posto anche l'attenzione sulle difficoltà riscontrate nella propria realtà, cosa che immagino si ripeterà anche nell'odierno dibattito. Perché, vedete, se c'è una cosa che è presente in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, questa è sicuramente la drammatica situazione delle carceri; non i dati sulla scuola, non i dati sull'occupazione, non i Non ci sono invece distinzioni tra le Regioni italiche rispetto al sovraffollamento, alla fatiscenza degli edifici, alla cronica carenza di personale, quello della polizia penitenziaria, ma anche del personale amministrativo, ed in particolare l'assoluta inadeguatezza della presenza degli assistenti sociali, degli psicologi e degli educatori. I tagli operati in questi anni al settore della giustizia stanno inoltre causando difficoltà di gestione e di efficienza amministrativa in tutti gli istituti penitenziari, causando in taluni casi una vera e propria "emergenza umanitaria". la si può vedere e toccare con mano; basti pensare alle condizioni di vita disumane in cui sono costretti a vivere i detenuti e che ha come conseguenza principale il costante aumento dei suicidi, dei tentati suicidi, degli atti di autolesionismo, di violenze e maltrattamenti, di aggressioni ad agenti di polizia penitenziaria, di rivolte. Sono tutti segnali di un malessere generalizzato che è oramai arrivato ad un punto di non ritorno.

Vede, signor Ministro, qualcuno si era illuso che il Governo, approvando il decreto del 13 gennaio 2010 che dichiarava lo stato di emergenza degli istituti penitenziari italiani, avesse preso finalmente coscienza della gravità del problema ed avrebbe agito di conseguenza, Invece poco si è mosso, anzi alcuni recenti provvedimenti legislativi hanno contribuito ad aumentare il numero dei carcerati. Dove sono finite le proposte di utilizzo delle caserme dismesse, i fantasiosi progetti per le carceri navigabili? E dov'è finito il piano straordinario per l'assunzione di 2.000 agenti? Passo ad illustrare alcuni dati che riguardano la mia Regione, il Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare la mia Provincia, Trieste: a luglio di quest'anno la Regione era al sesto posto nella graduatoria delle Regioni Regioni per quanto riguarda il sovraffollamento con una percentuale di 67,9 per cento; nel carcere di Tolmezzo, carcere di massima sicurezza, ci sono quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti disponibili. Nemmeno Udine e Pordenone stanno molto meglio. Attualmente a Trieste il numero dei carcerati è il più alto in assoluto dal dopoguerra ad oggi:

Causa il sovraffollamento e la mancanza di letti, 16 detenuti sono costretti a dormire sui materassi gettati a terra. Per non parlare poi delle difficoltà derivanti dalla presenza di un numero elevato di stranieri

Come ha detto recentemente il direttore del carcere, dottor Enrico Sbriglia, che è anche segretario nazionale del SI.DI.PE: "la situazione non è stata mai così critica". Dopo anni di dibattito c'è la totale incertezza sul futuro della casa circondariale di Gorizia, struttura obsoleta e completamente degradata. Non so quali risposte abbia ricevuto il sindaco Romoli che in questi giorni avrebbe dovuto incontrarla: il carcere

una storia infinita, nonostante vi siano disponibilità per la sua locazione. Ma oramai le parole si sprecano, i dati sono sotto gli occhi di tutti; voglio solo ribadire che abbiamo oltrepassato le misure di decenza, il che non è degno di un Paese civile, democratico; lo testimoniano i 34 suicidi nel primo semestre di quest'anno, ed i 532 tentati suicidi. Cito solo alcune proposte che potrebbero portare alla soluzione dei problemi: garantire ai detenuti il rispetto dei loro diritti fondamentali quali il lavoro, la salute, la formazione ed il reinserimento sociale. alle misure alternative, vorrei ricordare gli istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti, centri di accoglienza civili per gli immigrati, detenzione domiciliare per i reati di minore gravità. di una questione che va affrontata nell'ambito di una rivisitazione del sistema giustizia con una vera azione riformatrice. Ci sono due interventi che potrebbero essere l'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e le creazione delle condizioni affinché le madri con figli sotto i tre armi possano scontare la pena in un luogo diverso dal carcere. In conclusione, come cittadini penso dobbiamo indignarci per quello che sta succedendo nelle nostre carceri: guai a noi se dovessimo assuefarci anche a questo totale disprezzo per la vita umana. come classe politica, dobbiamo assumerci la responsabilità per trovare le soluzioni più appropriate. Chiedo pertanto anche al Governo di fare la propria parte, perché su questo tema ormai non ci sono p tempi supplementari.

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, l'ultimo provvedimento di amnistia risale al 1990.

di due terzi, articolo per articolo, l'amnistia si è fatta un obiettivo irraggiungibile in termini di parlamentarismo. Ecco la storia del nostro sistema, ferme restando le considerazioni di carattere generale che ha fatto stamattina il Ministro e che non ho difficoltà a condividere. furono sufficienti a non sfidare la simpatia e l'amicizia del mio presidente di Gruppo, senatore Gasparri, anticipando addirittura la collega Bernardini alla Camera, con un disegno di legge

che mi sono estranei. Ne ho difficoltà ad accedere, se maturerà nel dibattito, alla proposta anticipata dalla collega Bonino nel primo intervento di stamattina. Resta il fatto che, però, il sistema da vent'anni è cambiato. Siamo passati da legislature che vivevano di cronache di almeno un'amnistia annunciata a cronache di legislature, nelle quali il provvedimento di amnistia è *ecclesia pressa*. [**Presidenza

per affrontare una questione che è antica ed è moderna. Quando parlava stamattina il Ministro ho pensato con qualche orgoglio di senatore che gran parte dei suoi dati e delle sue considerazioni sono già in un bel volume del 2006, edito dal Senato, che raccoglie le ispezioni in merito al funzionamento del nostro sistema penitenziario, che nella XIV legislatura, il senatore Caruso ed il senatore Borea, rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione giustizia, avevano

che i detenuti in custodia cautelare sono più del 40 per cento. Ed allora dobbiamo avere abbastanza virilità nel prendere atto

è irrigidito, elasticizzato, alzando e abbassando tutti i possibili paletti, ma non ci siamo mai riusciti: Abbiamo scassato il codice, ma siamo ancora, signor Ministro, prigionieri 40 per cento che, conoscendo i suoi sentimenti, angoscia lei quanto i colleghi radicali e quanto altri in questa Aula. voglio partire proprio da una considerazione che ho avuto la fortuna di ascoltare il 28 luglio nel convegno del Senato in un intervento di Marco Pannella, meno alluvionale del solito e più nitido. Pannella indicava nell'ipocrisia, nel fallimento e nella catastrofe del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale il punto di degenerazione della giustizia. Non a caso

Se il nostro sistema di giustizia ci ha fatto quotidianamente rassegnare - le cronache sui giornali sono note - al ricatto quasi sempre, alla tortura molto spesso e molto spesso anche alla disumanità e alla viltà, vuol dire che noi questo principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è tempo che lo abbandoniamo. Da questo punto di vista il predecessore del Ministro, insieme al Governo, ha varato una riforma in gran parte costituzionale della giustizia che non entusiasma il collega Perduca il quale però forse è entusiasmato ancor meno dal clima di veto a discutere in cui si trascinano i lavori parlamentari da quando quel testo è stato presentato. 62 direi che dal punto di vista della storia del Parlamento è bene che il dibattito abbia per oggetto un tema come il pianeta carceri. Oggi, Oggi, che con tanta volgarità si dice che l'immunità parlamentare sarebbe un privilegio del singolo deputato cancellando tre secoli di storia del costituzionalismo e parlamentarismo inglese, parlamentarismo e carcere hanno una continuità e contiguità anche nella più domestica storia d'Italia. Penso a Filippo Turati, ai suoi discorsi sulla condizione delle carceri definite

doveroso un giro per Poggioreale. Signor Presidente, ho avuto dal personale un dato che mi indigna e mi umilia. Molti colleghi hanno parlato del lavoro nelle carceri e del lavoro utile. Ne parla la Costituzione, ma i lavori socialmente utili

Sono 30 anni che nella mia città denunzio il fatto che i disoccupati organizzati siano più organizzati che disoccupati. Avevo pensato

Anche per le 180.000 prescrizioni di cui ha parlato stamattina la collega Bonino e che costituiscono, di fatto, un'amnistia annuale alla quale siamo ormai rassegnati. Visto che il mio tempo è concluso, signor Presidente, ed in omaggio alle virtù del bicameralismo, vorrei segnalare quello che ho riscontrato l'altro ieri mattina al carcere di Poggioreale. C'è un detenuto, che è un parlamentare e che conserva tutte le sue prerogative, che non sono *ad personam*, sono dell'istituto costituzionale "Parlamento". Perché una magistratura, che non si vergogna di pensare all'ipotesi di accompagnamento coatto di un testimone, ha mancato da due mesi al suo dovere di procedere all'accompagnamento coatto alle sedute di Aula e di Commissione di questo parlamentare? Sono argomenti che non mi sembrano estranei a quello di stamattina. La ringrazio di avermi dato modo di esprimerli.

sento la eccezionalità della scelta dell'Assemblea del Senato di affrontare la questione delle carceri e sento la gravità delle ore che stiamo vivendo. L'allarme per l'Italia è altissimo: crolla con le Borse la fiducia; la vita di tante persone nel nostro Paese si è fatta incerta e difficile; la politica e il Governo sono messi alla prova senza più sconti, senza più tempo; sanzioni economiche e sanzioni politiche ci incalzano. Che cosa significa dunque in queste drammatiche ore questo dibattito sulle carceri del nostro Paese? Una parentesi tra incombenze più gravi? Il sussulto di un Parlamento sotto schiaffo e troppo a lungo distratto che ha deciso finalmente di non voltarsi dall'altra parte, di non passare oltre di fronte a luoghi dove vivono migliaia di persone, ai limiti della vivibilità, ai margini della città e della società? Potremo mai intervenire con efficacia, colleghi? L'interrogativo sembra evocare uno sforzo titanico. Eppure l'esito di questo dibattito non può non essere costituito da una decisione comune per cambiare le cose. Dentro il dramma dell'Italia c'è il dramma di questa realtà non più sopportabile, dentro l'emergenza dell'Italia c'è l'emergenza delle carceri. E l'iniziativa del Parlamento su sollecitazione dei Radicali questo significa oggi: affrontare subito il problema con tenace volontà per determinare il cambiamento necessario e possibile. Signor Ministro, lei sa, e lo ha anche detto: interventi concreti si possono fare da oggi, oltre l'ottima citazione delle parole del Presidente della Repubblica. Nelle vicende di questi giorni, così intrecciate, la nostra coscienza è una, le nostre responsabilità non sono separate, così come i diritti delle persone sono indivisibili, attraversano tutti i luoghi: nella civiltà di un popolo tutto si tiene. La Costituzione continua ad essere di fronte a noi come un vincolo imperativo già citato articolo 27). In realtà, tutta intera la Costituzione ci parla della persona, del diritto, dell'equilibrio in una società democratica, della sicurezza di una società democratica. Troppo a lungo abbiamo disatteso la Carta costituzionale, che è la bussola della vita, del diritto, dell'umanità, a casa nostra. Parecchie volte ho varcato, come altri colleghi, la soglia di un carcere con un senso di impotenza che oggi vorrei fosse almeno incrinato. Chi sta in carcere? Chi è recluso fino a un sovraffollamento intollerabile? Cittadini in attesa di giudizio, molti; tossicodipendenti, tanti; immigrati, in numero crescente; cittadini in espiazione della pena. Se vi possono essere misure alternative al carcere e se si può pensare la reclusione come *extrema ratio*, questo è il momento, modificando anche norme che si sono rivelate ottuse e inefficaci, come la legge Bossi-Fini e la legge Giovanardi-Fini. Se vi può essere, come vi è, un reinserimento controllato e vigilato nella vita sociale, questo è il momento di determinarlo. Nel carcere vivono migliaia di persone a cui sono negati i diritti costituzionali, senza i quali la vita non è vita, ed è a rischio, come il numero crescente di suicidi dimostra: detenuti esposti ogni momento alla violenza. Il diritto alla salute innanzi tutto. Il decreto del 1° aprile 2008 ha trasferito al Servizio sanitario nazionale la competenza in materia oltre le mura del carcere; occorre uno sforzo concertato perché questo passaggio sia effettivo in ogni Regione e in ogni territorio. Il Governo e la Conferenza Stato-Regioni ne discutano e diano l'impulso che ci si attende: vogliamo vedere risultati. Con la Commissione di inchiesta del Senato sul Servizio sanitario nazionale, come ha già riferito il presidente Marino, abbiamo preso in esame la vicenda di Stefano Cucchi. Ho curato la relazione finale insieme al collega Galioto, nella quale sono indicati i problemi, le responsabilità, le soluzioni; la magistratura sta facendo la sua parte. Un quadro di inadeguatezze, di paratie, di omertà è emerso e rappresenta il sistema carcerario di fronte alla salute, dentro il quale si può morire. Abbiamo anche affrontato la situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari e approvato all'unanimità la relazione finale che ne stabilisce il superamento. Come si vede, un pezzo di strada non piccolo è già stato compiuto; servono ora decisioni per superare ogni ostacolo. Ho visto, signor Ministro, nelle carceri il bisogno non soddisfatto di lavoro dentro e fuori le mura; il lavoro, che è elemento fondamentale della vita quotidiana per esprimersi, per avere relazioni, per avere dignità. Perché è così difficile, pur nelle condizioni giuridiche che lo consentono, renderlo praticabile? Si dirà che oggi manca il lavoro a molti fuori dal carcere. Io dico che questa è l'Italia di oggi e noi dobbiamo ripartire da qui, altrimenti sprofonderemo ancora di più e dovremo ricostruire il Paese da livelli ancora più bassi. un grande bisogno di istruzione e di formazione: dall'alfabetizzazione alla possibile frequenza a distanza dell'università. Vi sono esperienze positive, ma occorre fare molto di più. Quale posto occupa il Ministero dell'istruzione in questo settore? Certo, se è in abbandono l'intero sistema di istruzione figuriamoci l'intervento nelle carceri: i tagli sono arrivati anche lì, puntualissimi; eppure, la conoscenza è la strada maestra per affrontare la detenzione. Salute, lavoro, scuola: è chiamata in causa non solo l'amministrazione penitenziaria, non solo i Ministeri interessati ma il territorio, i sindaci, le Province, le Regioni, le ASL. Il carcere dentro una rete. Conosco la realtà di Parma, di Reggio Emilia e dell'Emilia-Romagna e il lavoro delle istituzioni e del volontariato: una goccia nel mare, ma la strada è tracciata. È possibile aprire spazi di vita e di dignità:

in condizioni di disagio insostenibili. Il Governo intervenga con l'assegnazione del personale necessario, degli educatori e degli psicologi, senza i quali i progetti personalizzati non sono possibili. Vi sono detenuti malati che chiedono di essere trasferiti vicino ai familiari, e la burocrazia spesso li dimentica. A tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute si è istituita, a tutti i livelli, la figura del Garante: è il minimo che si possa fare per fare delle carceri un luogo dove abiti il diritto e, proprio per questo, strumento certo di giustizia e di sicurezza per la società. Signor Presidente, la società italiana è più avanti di noi: diverse associazioni, giuristi e sindacati ci hanno sollecitato, con un documento comune ricco di proposte, a intervenire. L'impegno del Senato oggi e della Camera domani non può rimanere una dichiarazione di intenti: sarebbe colpevole. Si deve agire: lo faccia il Governo e lo facciano le istituzioni che ne hanno competenza. Diamoci un tempo, anche più lungo nella riflessione, come richiesto dalla senatrice Bonino, senatrice Bonino, e tra sei mesi verifichiamo in quest'Aula lo stato delle cose, qualunque cosa succeda. Più grande è l'emergenza, più grande in questo istante e in ogni istante è la nostra responsabilità, perché l'Italia non smetterà di essere Italia e le nostre responsabilità continueranno ad inchiodarci al dovere di attuare la Carta costituzionale in ogni spazio della società italiana, anche con una crescita bloccata e una politica senza orizzonte. Per quanto delegittimato nell'opinione pubblica, il Parlamento non si può dimettere dalle sue prerogative e dalle sue responsabilità, e là dove l'uomo è più offeso nella sua dignità, come nelle carceri, là è necessario e urgente che questa dignità sia riportata. Là dove il diritto non è realizzato, lo Stato di diritto deve essere presente, perché anche lì vive la Repubblica e vive l'Europa, con il suo presidio sul diritto, sul confine tra civiltà e barbarie: non paghino ancora una volta gli ultimi questo tempo duro e senza certezze dell'Italia!

signor Ministro, signora Sottosegretario, cari colleghi, il 24 dicembre 2010, la vigilia di Natale, sono andata in visita al carcere di Lucca insieme al senatore Marcucci per portare i consueti auguri, ma mentre varcavo quel portone, quei cancelli scrostati e arrugginiti, sentivo nel cuore un profondo disagio, un imbarazzo della coscienza che si dibatteva tra il desiderio di portare una parola di conforto e il senso di impotenza di fronte a una situazione carceraria insostenibile, ignobile, tanto più per una città molto cattolica come quella di Lucca. Forse per questa inquietudine, forse per i tristi pensieri e la mia distrazione, nel pavimento sconnesso del chiostro ho lasciato per sempre la piena funzionalità del mio piede sinistro, toccando con mano, anzi con il piede, la fatiscenza, il degrado e la pericolosità dell'edificio. Ciononostante ci sono tornata a Ferragosto con la speranza che le interrogazioni presentate, gli interventi sulla stampa, gli appelli al Governo avessero prodotto qualche effetto ma, ahimè, la situazione non era affatto migliorata: il direttore si era ritrovato sulle spalle la direzione di altre due carceri, quella di Pistoia e quella di Prato; il personale in organico era ridotto al 40 per cento di quello previsto; i detenuti erano 175, a fronte di una capienza di 99; meno, molto meno di 3 metri quadrati per detenuto; attività di recupero e socializzazione zero. Ma questa è solo una piccola testimonianza di una situazione carceraria che è drammatica, indegna di una potenza occidentale che siede ai maggiori tavoli internazionali e che ha una storia cosi radicata di civiltà giuridica democratica. I dati che lei ci ha fornito, signor Ministro, sono allarmanti. Li conoscevamo, ma così certificati pesano ancora di più. Il dato più sconcertante riguarda l'affollamento. Lei ci ha riferito che in un sistema carcerario che potrebbe ospitare 45.732 detenuti, Sono aumentati, è vero, gli ingressi di detenuti stranieri, probabilmente a causa della propensione all'arresto anche nei casi in cui si deve semplicemente procedere all'identificazione. Ma non è tutto: 12.000 persone in attesa di giudizio. Veniamo ai costi. Secondo un rapporto di Antigone, associazione che si interessa di giustizia penale, per ogni detenuto si spendono 157 euro al giorno. Di questi, solo 8 euro sono destinati al vitto e alla salute; il resto sono spese che riguardano manutenzione dei fabbricati, gestione ordinaria e personale, con un preoccupante taglio alle risorse impiegate proprio per la sanità nelle carceri. Viene da chiedersi: quanto si risparmierebbe se venissero aumentate le pene alternative? E, soprattutto, quanto ne guadagnerebbero i detenuti in termini di qualità della vita? Quindi, sovraffollamento, spazi assolutamente insufficienti, degrado delle strutture, carenze di servizi e di personale (lei ci ha detto che mancano ben 5.877 unità)

Il diritto alla salute dei detenuti è rimasto sulla carta. Dopo l'assegnazione dell'assistenza sanitaria in carcere alle ASL (Sicilia esclusa), che non hanno né i mezzi, né le conoscenze necessarie, né la progettazione giusta per operare nei luoghi di restrizione della libertà,

Sia ben chiaro: il carcere non può essere un piacevole luogo di soggiorno gestito a spese dei contribuenti. Sottolineo questo aspetto per contrastare quella becera e gretta propaganda - tutta ideologica propria di una certa cultura che non vuol ricordare tutte quelle conquiste civili divenute patrimonio fondante della nostra Costituzione, dove - lo ricordo - all'articolo 27 si legge: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il carcere dovrebbe dunque essere il luogo dove, una volta condannati, si sconta una pena, si paga (con umanità) un debito con la società, si rieduca, ma paradossalmente oggi nelle carceri italiane, nella situazione attuale, a spese dei contribuenti e della loro sicurezza, si creano e formano le nuove leve della Signor Ministro, come si può non capire che questo stato di cose è un vero generatore di ulteriore illegalità? Chiudere gli occhi è un errore. Occorre investire sul sistema carcerario, ma con progetti seri, che non restino sulla carta, come il piano di potenziamento dell'edilizia carceraria e l'adeguamento dell'organico della Polizia penitenziaria. Servono strutture intermedie, come lei ha ricordato stamani, ma soprattutto un forte investimento in risorse umane, in operatori specializzati in grado di costruire percorsi di Non so se un provvedimento di clemenza come l'amnistia sia la soluzione più giusta. Del resto, come ci ricordava la senatrice Emma Bonino, siamo di fronte Di sicuro però so che il sistema carcerario attuale, oltre a mettere fuori legge lo Stato italiano, condannato addirittura dalla Commissione europea per violazione con riferimento al reato di tortura (oltre 1.000 condanne), serve solo a privare della libertà e spesso dei diritti umani più elementari chi deve scontare una pena, non rieduca nessuno, anzi è spesso il maggior fornitore di manodopera per la malavita organizzata. Capisco che il problema è difficile, ma il Governo una volta tanto deve andare oltre l'emergenza, pensare a una riforma strutturale che da un lato assicuri il corretto e civile trattamento dei detenuti e dall'altro dia vita a un sistema giudiziario penale funzionante che assicuri l'effettività dalla sanzione ma anche il reinserimento reinserimento e che soprattutto risponda all'esigenza di sicurezza che la società esprime. Occorre una stagione di sereno confronto tra le forze politiche, un dibattito serio e aperto nella società civile, che porti a una radicale soluzione del problema, che renda credibilità al nostro Paese e soprattutto ci restituisca quel senso di umanità previsto dalla Costituzione e al quale ci richiama continuamente anche il nostro Presidente della Repubblica, ma soprattutto, mi auguro, la nostra coscienza.

inoltre che la gravità di questa convocazione debba farci esaminare con calma quei numeri, quei dati e quelle cifre, certo senso si è interrotto nella fase che forse poteva essere più interessante. Quei numeri, quelle cifre, quella realtà, quella situazione di completa e assoluta illegalità in qualche modo va interrotta.

per dare aria a un sistema che non ne aveva e che oggi potrebbero essere viste come delle misure tampone, provvisorie, di cui discutere solo in questo senso, appunto come misure tampone. Ma cosa ci potrebbe essere di più strutturale se non eliminare il sovraffollamento dei processi pendenti sui pendenti sui tavoli e nelle aule dei nostri tribunali? Cosa ci potrebbe essere di più strutturale che ridurre da

per far ripartire la macchina di un sistema giudiziario che evidentemente è bloccato e produce i risultati illustrati

anche degli italiani che sono nelle carceri italiane e, come punta massima della discarica sociale del sistema penitenziario, ci sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, la discarica delle discariche, con le persone che nessuno vuole assolutamente È la malattia che viene incarcerata; è il disagio psichiatrico di quella persona che viene messo dietro le sbarre,

la punta dell'*iceberg* del sistema penitenziario. Allora, di fronte alla gravità della convocazione di oggi, alla gravità dei dati che ci ha fornito e che continuiamo ad elencare nei vari interventi,

È qui che lei si è interrotto, auspicando un sereno confronto. Ma il sereno confronto parte anche dalle proposte, dalla responsabilità

ma è obbligatorio. In caso contrario, non possiamo fare altro che prendere atto che siamo in una situazione di completa illegalità. Se però si prende atto che l'illegalità viene certificata dal Presidente della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dal Governo e dal Ministro della giustizia, a un certo punto questa illegalità andrà interrotta, altrimenti è tutto illegale, anche la stessa certificazione dell'illegalità.

ha iniziato ieri, e da una settimana è in sciopero della fame. E io credo che sia utile leggervi base ai quali Marco Pannella ritiene l'amnistia un atto dovuto, un atto obbligato, un atto che non è un tampone per bloccare qualcosa ma è «L'amnistia non solamente interromperebbe la flagranza di un comportamento assolutamente criminale dello Stato partitocratico in concreto, contro lo Stato di Diritto la Repubblica democratica, contro centinaia e centinaia di migliaia - anzi di milioni - di persone. In sintesi contro i Diritti Umani, con responsabilità che dovrebbero essere giudicate e condannate dalla Corte Penale Internazionale (e a questo fine dobbiamo preparare urgentemente la relativa, documentatissima, urgentissima denuncia, individuando gli strumenti e le modalità tecniche atte a farli ricevere); non solamente costituirebbe il solo provvedimento atto ad avviare in modo irreversibile da subito» - sottolinea da subito - «il processo di riforma della Giustizia, del Regime partitocratico, sovraffollata e disastrata

sua liberazione dal nazifascismo ma non da ogni altra illusoria, mortale utopia che ha reso tragico il secolo precedente, e già ipoteca del secolo che viviamo

i criminali sono già fuori. Non è quello il problema. La nostra proposta è quella dell'amnistia. Avanzatene altre. Proponete qualsiasi altra cosa, ma non limitiamoci oggi ad elencare il disastro del sistema penitenziario.

ho apprezzato la radiografia da lei fatta dell'attuale situazione e i dati che ci ha fornito. fornito. Mi sarei aspettato che venisse toccato qualche punto un po' caldo, del quale lei non porta nessuna responsabilità, che però forse è il caso di affrontare. Vorrei partire da quello che nel giugno del 2008 il ministro Alfano disse al Parlamento nel prospettare le soluzioni per il problema carcere. diede quattro indicazioni molto precise: parlò necessità di creare i circuiti differenziati, che non so se ora coincide con la sua idea delle carceri a bassa sicurezza; parlò dei trattati internazionali per la consegna, ai Paesi d'origine, dei detenuti in in esecuzione; parlò della costruzione dei padiglioni all'interno degli istituti già esistenti; e poi parlò del braccialetto elettronico.

nel senso che Paesi di origine della popolazione carceraria estera non stipulano trattati. Peraltro, c'è un ulteriore aspetto che è stato evidenziato nel corso dei dibattiti che si sono svolti su questo tema: la consegna dei detenuti stranieri ai Paesi d'origine comporterebbe, in applicazione del principio di reciprocità, che noi prendessimo in carico gli italiani che sono detenuti all'estero,

non si fanno trattati. I braccialetti elettronici rimangono uno strano e misterioso argomento, che peraltro è costato, e continua a costare - fino a quest'anno,

siamo arrivati al 2011, abbiamo pagato 11 milioni di euro l'anno. Possibile che non si sia perfezionato il sistema e non si sia trovato il modo di sganciarsi dal contratto? Abbiamo regalato a Telecom 110 milioni: perché?

Indubbiamente questa situazione ci deve far riflettere sull'istituto della custodia cautelare (la risposta che si è data negli ultimi tempi è stata quella di ridisegnare in maniera più appesantita cioè si è ampliata la platea di esclusione del carcere come misura residuale: la politica è andata in questa direzione), come risposta immediata a un bisogno di sicurezza della collettività. In pratica, dato che non si riesce a fare il processo, si risponde immediatamente al bisogno di sicurezza dicendo

risposta, questa. Due anni fa venne introdotto il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel nostro Paese,

ucciderebbe definitivamente il sistema penale. Si propone poi l'amnistia. Francamente non riesco a cogliere il nesso

l'amnistia con il carcere, a meno che non si dica che, applicando l'amnistia, liberiamo le scrivanie (usando un modo di dire). Con l'indulto si svuota il carcere, con l'amnistia si svuotano i cassetti:

l'eliminazione del processo agli irreperibili, che sono decine di migliaia,

la depenalizzazione dei reati di fascia bassa; e ancora, l'introduzione di quell'istituto che ha funzionato e funziona per i minori, bassa, l'istituto dell'affidamento in prova, non sul giudizio non sul giudizio definitivo: anticipare l'istituto dell'affidamento in prova pattizia prima del giudizio, cioè non dopo i tre gradi, ma proponendo all'imputato di un reato di fascia bassa un affidamento in prova, determinerebbe lo stesso risultato dell'affidamento in prova

avanzato sin dal giugno 2008, ma non si è aperto nessun dibattito. Purtroppo, abbiamo perso oltre tre anni, con una situazione carceraria che non può essere disgiunta

della macchina che non funziona; né possiamo risolverlo con provvedimenti tampone che non risolverebbero per nulla il problema, mentre le soluzioni ci sono.

quelle di riformare il codice penale e la procedura introducendo anche determinati istituti nuovi e riesaminando - ma ci vorrà un dibattito in proposito

Presidente, Ministro, abbiamo ascoltato la sua relazione di questa mattina. Mi permetterei di definirla come una relazione che non ha nascosto nessun profilo e nessun aspetto del problema. Quindi non è una lettura clemente. una lettura clemente. Lei ha usato espressioni pesanti, come si addicono ad una realtà che è dinanzi ai nostri occhi, la cui gravità è stata segnalata dentro e fuori dal Paese da fonti autorevoli, ad esempio, dalla Corte di giustizia. Anche il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dover fare un richiamo forte affinché il Parlamento ed il Governo si occupassero di una situazione drammatica, che coglie ancora una volta un aspetto importante della cittadinanza in questo Paese, seppure limitata e condizionata, come è nei limiti di libertà che il carcere impone, al cittadino che si è macchiato di un reato. Ma la condizione è insostenibile. Siamo cioè lontanissimi dall'articolo 27 della Costituzione,

siamo proprio fuori dal rispetto della dignità dell'uomo nella sua condizione di carcerato. E noi non possiamo permettercelo perché,

per il suo sistema carcerario, ne avremmo e ne abbiamo quel giudizio anche di meraviglia. Quindi, la sua è un'analisi che non ha nascosto questi aspetti, ma, se mi consente, Ministro, manca di una proposta. Si è mosso il Parlamento, e questo ramo del Parlamento ha visto, sull'*input* dell'apprezzabilissima e condivisibile iniziativa della presidente Bonino, 141 senatori che hanno ritenuto di di dare sostegno all'iniziativa di questa mattina. Ma non può e non deve accadere - e credo che non sia neanche nei suoi auspici

da qui ad un tempo ben definito, di quel numero esageratissimo di popolazione carceraria di 67.000 unità, in rapporto alla capienza di 42.000 unità.

Naturalmente, anche nelle analisi ci può essere una diversa valutazione. Molti di noi sono convinti che la scarsa attenzione alle autentiche e vere riforme di cui il sistema giudiziario aveva bisogno si riflette anche da molto tempo sul sistema carcerario.

giustizia lenta e quindi ad un approdo alle sentenze e alle condanne in un tempo lunghissimo rispetto al bisogno di sicurezza che la comunità aveva, ha introdotto norme che hanno esaltato e ingigantito la carcerazione preventiva, e così abbiamo naturalmente risposto in maniera anomala rispetto ad una soluzione ordinaria. ordinaria. Non sarebbe neppure tanto strumentale se dicessi, come qualche volta mi è capitato, che tre anni e qualche mese sono stati sprecati per altri aspetti della giustizia e non per il cuore delle sue questioni, che richiedevano riti più veloci, procedure più snelle, informatizzazione del settore in più. Il percorso ci porta molto lontano. Le analisi sono importanti perché fanno prendere bene e coerentemente le decisioni, ma qui noi dobbiamo concludere con un'operazione che sia più circoscritta, più determinata e definita. Vi sono punti sui quali c'è una convergenza: c'è una convergenza: qualche ritocco al sistema normativo che prevede la carcerazione preventiva, a mio avviso, va messo in campo. Le pene alternative vanno rafforzate e devono essere devono essere più robuste; la depenalizzazione è un altro tema in campo. I due grandi filoni che alimentano

concludo il mio intervento con una convinzione molto forte e con un giudizio di insoddisfazione: è cruda l'analisi ma è debolissimo l'approdo, è debolissimo l'approdo, perché d'accordo che è in corso il piano di ampliamento delle strutture carcerarie, ma tra le risposte è una la risposta, e non può essere la prima; ne conveniamo tutti, e anche lei, nella parte terminale dell'intervento, lo ha sottolineato. È un piano che peraltro meriterebbe, Ministro, una più puntuale e dettagliata informazione, perché anche noi in Commissione giustizia abbiamo pochi elementi per sapere come si sviluppa, come sta andando e se questa promessa di completamento

tradurre la volontà di ridurre questa patologia mediante un pacchetto definito di proposte, e in tempi brevissimi.

di cui alcuni colleghi hanno già trattato, per la puntualità di alcuni dati che sono stati estrapolati, che consentono quindi, nella discussione di oggi e in quella che ne verrà, un'analisi

condivisa se possibile, a mettere in campo alcune azioni per dare una soluzione ai problemi che sono stati prospettati stamattina. Tra questi credo vi sia anche la domanda cui siamo tenuti a dare una risposta, e che è stata oggetto anche di alcuni interventi: vi è la possibile reiterazione di un altro provvedimento che, oltre a estinguere la pena, possa andare anche nella direzione di estinguere il reato?

ma anche perché è stato detto che vengono prescritti 180.000 processi penali, che noi riteniamo che questo sia il fallimento dello Stato, al di là dei motivi e delle misure

essere un Paese in cui c'è la prescrizione breve nel processo lungo, per cui non si arriva a decidere se un cittadino sia innocente o colpevole; qualora sia stato invece condannato non si è in grado

molto lunga, di oggi (credo anche positiva, perché è stata una sollecitazione giusta) avrà un senso se riusciremo ad affidare alla Commissione

in questo caso di amnistia, che è stato peraltro anche ben spiegato e ben articolato, ma bisogna anche far sì che vengano risolte ed eliminate in radice le condizioni che poi portano all'emergenza.

La descrizione è stata fatta, e non la ripeto. Il problema delle strutture: il piano carceri prevedeva 47 nuovi padiglioni, 11 nuovi istituti, 600 milioni di euro di investimenti entro il 2012. Ebbene, mi pare che siamo molto in ritardo.

In questo modo, credo che saremo in grado di fare in maniera che la pena non sia ulteriormente afflittiva. La pena prevista è la sottrazione della libertà: non è la mancanza di assistenza sanitaria, il sovraffollamento, vivere in spazi ristretti, non è la mancanza assoluta della possibilità di esercitare una qualche forma di lavoro. Noi avevamo presentato anche un disegno di legge che, per quanto riguarda le misure alternative, consentisse a chi deve scontare l'ultimo anno di detenzione domiciliare la possibilità di farlo lavorando presso una ONLUS.

il trattamento e la situazione carceraria possono dimostrare l'efficacia e l'efficienza di uno Stato, ma devono dare anche le cifra del suo senso di civiltà e di rispetto dei diritti umani. *(Applausi

Presidente, signor Ministro, colleghi, bene hanno fatto i colleghi radicali a prendere l'iniziativa, cui molti di noi hanno aderito, di impegnare l'Aula in queste sedute

delle condizioni in cui vivono oggi i detenuti, scarto di cui ha parlato autorevolmente, molto meglio di quanto possa farlo io, il Presidente della Repubblica, che anche il Ministro ha voluto

che possiamo svolgere in questa nostra giornata si concluda con risposte assolutamente vaghe e inadeguate, dico subito che condivido la proposta della senatrice Bonino di prenderci tutto il tempo necessario affinché a questa

i dati sul sovraffollamento che lei ha voluto dare sono quelli noti; l'unico che non ho ben capito, e che stride un poco con la concretezza dell'esperienza di chi di noi è andato nelle carceri, è quello secondo il quale

Così non è, evidentemente, in molti dei nostri istituti penitenziari, la cui situazione è veramente grave. Tra i molti sintomi di disagio, il più grave è sicuramente quello delle morti che avvengono in carcere e, tra quelle, dei suicidi. Vincenzo Lemmo, Loredana Berlingeri, Carlo Saturno, 'Mehedi Kadi, Moez Atadi: sono i nomi di alcuni soltanto dei 1.890 detenuti morti, di cui 673 suicidi, nelle carceri italiane negli ultimi dieci anni.

che di queste donne e questi uomini, se non viene denunciato il decesso o il tentato suicidio dai parenti o dalle associazioni che meritoriamente si battono in difesa dei diritti dei detenuti, spesso nemmeno conosciamo il nome.

per liberare fino in fondo gli istituti penitenziari. Le misure alternative, di cui anche il Ministro ha parlato oggi, mi sembra siano

di considerare anche l'amnistia e l'indulto come strumenti da prendere in esame per risolvere il drammatico problema. Colleghi, sono tra coloro che nella scorsa legislatura hanno votato a e, forse contrariamente ad altri che lo votarono insieme a me, non sono affatto pentito di quel voto. So che nel 2006-2007, quando, per effetto dell'indulto, la popolazione detenuta era tornata nei limiti di capienza prevista per il sistema penitenziario, i detenuti morti furono il minimo

Ministro, su questi episodi ho presentato moltissime interrogazioni (credo siano 15) insieme a tanti altri colleghi, e mai il Governo ha risposto. Sarebbe forse opportuno che invece il Governo rispondesse ai parlamentari quando pongono problemi In conclusione del mio intervento, vorrei affrontare uno dei motivi principali per cui le carceri italiane sono giunte all'attuale situazione, tanto intollerabile, di sovraffollamento. Io credo che uno dei motivi principali - dobbiamo dirlo con chiarezza - sia quell'ingiusta ed inefficace legge che porta il nome del sottosegretario Giovanardi. Nel 2009, in occasione della Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope convocata dal sottosegretario Giovanardi, le associazioni «La società della ragione», «*Forum* Droghe» e «Antigone» presentarono a Trieste un Libro bianco sui primi tre anni di applicazione della legge punitiva del 2006. Ovviamente la Conferenza governativa eluse il confronto su quei dati, ma fece male, perché in quel Libro bianco del 2009 si evidenziavano gli effetti negativi dell'inasprimento dell'inasprimento penale che cominciavano ad emergere con chiarezza. Oggi dalla lettura del secondo Libro bianco emerge che non vi è alcun dubbio sui danni collaterali della legge antidroga, repressiva e criminogena,

Sono tante le iniziative che possiamo presentare: io ed il collega Della Seta, ad esempio, abbiamo presentato un disegno di legge che vuole rimediare a queste distorsioni. Qualche collega ci ha detto, giustamente,

carceraria. Forse, è un problema strutturale che va affrontato, poiché le carceri italiane sono vecchie fortezze dell'epoca borbonica o papalina.

hanno realizzato dei complessi nelle campagne dove i detenuti possono lavorare e vivere con maggiore libertà.

Creiamo un'edilizia carceraria nuova, piantiamola con le vecchie fortezze, con i vecchi castelli e cerchiamo di spostare tutto

Mettiamoci un po' di fantasia, cerchiamo di far sì che l'edilizia carceraria venga ripristinata in modo diverso, evitiamo di pensare che possiamo costruire nuove carceri: lo stato economico del Paese non lo consente. Non lo faremo, e cerchiamo di mettere un po' di fantasia su un modello nuovo. La fantasia nel governare è uno dei requisiti essenziali.

terzo comma, della nostra Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Al centro, come è evidente, rimane l'uomo, la persona, come risorsa fondamentale per la società, anche nelle condizioni di reclusione e di espiazione della pena. Il nostro Presidente della Repubblica, lo ha ricordato anche il Ministro nel suo intervento iniziale, recentemente ha parlato di uno Stato umiliato e di prepotente urgenza, riferendosi al sistema delle carceri italiano e al suo drammatico sovraffollamento. Un Paese - il nostro - che non garantisce talvolta neppure la dignità minima per le persone recluse, e che quindi non si può definire uno Stato democratico, e la nostra società non può dirsi civile. Persone costrette a convivere con letti a castello tripli in meno di 9 metri quadrati di cella e ad utilizzare lo spazio angusto della latrina anche come dispensa alimentare e angolo cottura per scaldare le vivande: queste sono le condizioni ordinarie della detenzione nel nostro Paese! Le sentenze di condanna non mancano, dalla sentenza della Corte europea del 2009 per il caso Sulejmanovic, rispetto al quale la Corte ha dichiarato il reato di tortura nei confronti del detenuto che non abbia a disposizione almeno tre metri quadrati di spazio nella cella. Nel caso specifico, Sulejmanovic era detenuto in una delle carceri meglio gestite e in cui si vive meglio in Italia, il carcere di Rebibbia, dove poteva contare su ben 2,7 metri quadrati. Ricordo che il parametro utilizzato dalla Corte europea dei diritti umani è, per ogni detenuto, di quattro metri quadrati in cella multipla e di sette metri quadrati in cella singola.

Complessivamente rappresentano oltre la metà della popolazione carceraria, se si considerano gli appellanti e i ricorrenti in Cassazione: detenuti che poi spesso escono per decorrenza dei termini o perché la condanna è inferiore alla carcerazione preventiva. Un'altra considerazione è poi relativa alla tassonomia della popolazione carceraria: almeno un terzo sono i tossicodipendenti o i detenuti per reati correlati allo spaccio di sostanze stupefacenti, (un dato, quello relativo alla penalizzazione delle droghe

Ricordiamoci però che sono quasi la metà quelli che negli Stati Uniti sono detenuti per questi motivi, ma intanto da noi la parte prevalente è detenzione sociale. Insomma, come al solito, la repressione finisce per orientarsi verso le fasce di marginalità: tossicodipendenti, extracomunitari e malati mentali. Sono i cosiddetti prodotti della Bossi-Fini, che criminalizza l'irregolarità amministrativa degli immigrati; della Fini-Giovanardi, che considera altamente criminale l'uso delle droghe leggere e della Cirielli, che infierisce sulla recidiva. Reati che andrebbero affrontati con soluzioni mediche o amministrative e rispetto ai quali la funzione rieducativa dovrebbe essere prioritaria. In compenso, invece, il numero dei suicidi è in aumento,

è costato alle casse dello Stato circa 29 miliardi di euro, di cui solo 11 centesimi al giorno per la rieducazione. Ma dove e come sono stati spesi gli oltre due miliardi e mezzo all'anno? Che cosa ci può dire Ministro - ad esempio - dei 110 milioni a Telecom, per un contratto decennale stipulato nel 2003, che ancora oggi garantisce una centrale operativa 24 ore su 24 per 400 braccialetti elettronici (i più cari d'Europa, super tecnologici e leggerissimi, meno di 50 grammi l'uno), di cui solo una decina sono però quelli effettivamente assegnati. Organi di stampa hanno annunciato che il nuovo piano carceri ha realizzato circa 2.000 posti (costruiti o ristrutturati) in tutta Italia, tutti, puntualmente, inutilizzati: il nuovo padiglione a Cuneo, 400 posti, ancora vuoto; a Velletri, 200 posti, ancora vuoti; una nuova ala realizzata nel carcere di Nuoro, ancora vuota; una nuova ala anche ad Avellino, ancora vuota; una nuovo padiglione nel carcere circondariale della mia città di Livorno, ancora vuoto; il carcere di Rieti ancora semivuoto, come i reparti di Enna e Barcellona Pozzo di Gotto; per non parlare del carcere di Gela, definito il carcere dei guardiani della luce: 48 celle senza detenuti, ma con personale che vi lavora ogni giorno che si limita ad accendere e spegnere l'illuminazione. Inoltre, vi sono molti, troppi, edifici nuovi e non (Pinerolo, San Valentino in Abruzzo, Monopoli ed altri), che non possono funzionare per la mancanza di operatori specializzati, come educatori, psicologi Lo stesso organico della Polizia penitenziaria è nei fatti abbandonato a se stesso con drammatici riduzioni di organico, talvolta stimati fino alla metà di quelli previsti dalle piante organiche. I disagi e i disservizi, ma soprattutto il livello della sicurezza che può essere garantita in condizioni di sovraffollamento, promiscuità, segregazione e casi multidiagnosi, sono facilmente immaginabili. un sistema che ha urgente bisogno di controlli, razionalizzazioni, ma non di tagli lineari, come è avvenuto nelle ultime finanziarie. L'unico taglio ammissibile è quello sui detenuti, ma questa volta non basterà un provvedimento di clemenza, indulto o amnistia che sia. Occorre piuttosto preventivamente pensare a misure che si occupino delle vere cause di un male ormai divenuto endemico per il nostro Paese. Bisogna ripensare agli illeciti penalizzati, che sono serviti più come strumento di propaganda che per arginare effettivamente i fenomeni criminali, che hanno portato in carcere persone che non sono realmente pericolose, lasciando fuori i ladri e i criminali veri. Insomma, per il sistema penitenziario italiano la ricetta giusta è nota: un piano d'interventi articolato e urgente, che va dalla depenalizzazione di molti reati al piano infrastrutturale delle carceri, dalla rieducazione, al funzionamento effettivo del braccialetto elettronico (come avviene normalmente negli altri Paesi), dall'ampliamento degli organici ad un sistema giudiziario che sia messo in grado di funzionare in tempi ragionevoli e certi. Come è evidente, un intero modello chiede di essere ripensato, mettendo al centro la persona, sia che sia reclusa o che vi operi per la sua custodia, utilizzandone al meglio le potenzialità e le motivazioni che non si esauriscono in quelle condizioni, ma che proprio da quelle possono trovare nuove energie e nuova utilità per la società. Il lavoro, anche in quelle condizioni, può costituire una straordinaria forma di riscatto e di educazione. Ci sono esperienze meravigliose e straordinarie - come lei sa, Ministro - che in questi anni si sono sviluppate grazie alla generosa sensibilità di molte associazioni di volontariato laiche e cattoliche, operanti nei nostri istituti penitenziari, talvolta perfino mal tollerate ed ostacolate dalle stesse strutture. Vanno invece valorizzate: accendiamo i riflettori su queste isole, facciamone un modello da perseguire. Rendiamo queste esperienze imprese sociali, di utilità sociale e di interesse generale, perché nessuna persona sia un rifiuto a perdere, per quanto male abbia potuto commettere. La nostra cultura cristiana ci suggerisce di perseguire il perdono piuttosto che la vendetta; ci stimola all'interesse e all'attenzione verso l'altro piuttosto che all'indifferenza. Facciamo allora in modo che anche questi giusti precetti non si smarriscano proprio nei luoghi dove di essi maggiore ve ne è il bisogno.

In Italia sono più di un milione le persone colpite dalla demenza, delle quali 800.000 sono malate di Alzheimer. Sono perciò 800.000 le famiglie italiane che chiedono attenzione per una patologia che, insieme al malato, condiziona pesantemente la vita dei familiari. *Alzheimer Disease International* lancia un appello perché tutti si ricordino delle persone colpite dalla malattia e mettano in atto comportamenti adeguati per aiutare chi soffre. Lo *slogan* di quest'anno offre due indicazioni forti. La prima riguarda chi si accosta ad un ammalato, sia questi un professionista della salute oppure un parente, un vicino di casa, un amico: la dignità umana e la nobiltà non scompaiono mai, il volto conserva i segni di una storia, seppure resi irriconoscibili dalla malattia. Anche la luce degli occhi sembra spenta, ma sono occhi che hanno visto, amato, trasmesso messaggi vitali per molti anni. Se guardiamo in faccia la persona colpita da una demenza, allontaniamo da noi il rischio di considerarla come un essere inanimato, di offrirle una cura generica. Una seconda indicazione riguarda soprattutto i medici, perché suggerisce che ogni persona malata di demenza è diversa da qualsiasi altra e che una medicina ben fatta impone di approfondire la conoscenza di ogni singolo; le storie sono diverse, i sintomi hanno gravità e durata diversi, la sofferenza del malato e della sua famiglia è assolutamente individuale. La cronicità di una malattia non delinea percorsi uguali. Infine, «I volti della demenza» davanti al nostro sguardo rappresentano uno stimolo continuo a migliorare le cure attraverso la ricerca scientifica, che porta trattamenti innovativi e al miglioramento delle metodologie di cura. A noi legislatori compete di ricordarsi nella programmazione sanitaria di questi bisogni essenziali. *(Applausi